del servizio di noleggio con conducente, cui risponderà il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Matteoli. Si fa presente che è in corso la diretta televisiva della RAI, che avrà la durata di un'ora e si esaurirà con i primi due argomenti.

Ministro, considerato che l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria è l'unica arteria di collegamento da e per la Calabria, la Sicilia e il resto d'Italia; considerato che, a seguito dei fenomeni di maltempo, è stata recentemente colpita da frane e smottamenti che hanno causato anche la morte di due persone e peggiorato lo stato di grave precarietà nel quale versa da decenni; considerato tra l'altro che il sottosegretario di Stato per la Protezione civile Bertolaso ha definito "totalmente inadeguata" la struttura calabrese per fronteggiare le emergenze e che ormai da tempo immemorabile tale arteria attende un completamento che renda più sicuro e regolare il traffico di merci e di persone; considerato, infine, che per superare le oggettive difficoltà occorrerebbe un coordinamento tra Ministero, ANAS, prefettura, Polizia stradale e Protezione civile, si chiede di sapere se risulti al Ministro un piano dell'ANAS finalizzato a garantire la sicurezza della circolazione stradale, gravemente compromessa, e la regolarità dei flussi di traffico turistico e commerciale di merci, mezzi e persone da e per la Calabria e la Sicilia, particolarmente importante alla vigilia, tra l'altro, della stagione primaverile ed estiva. chiede di sapere, inoltre, se l'eventuale predisposizione di questo piano sia stata fatta coinvolgendo tutte le autorità e, del caso, quali. *(PD)*. Signor Presidente, onorevole Ministro, il progetto di ammodernamento e messa in sicurezza dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria costituisce una priorità di assoluta valenza strategica nella politica infrastrutturale del Paese;

idrogeologici sulla Salerno-Reggio Calabria; è stato proprio uno smottamento a causare il crollo di un muro di sostegno sulla carreggiata sud, nei pressi dello svincolo di Rogliano-Grimaldi, la notte del 25 gennaio 2009, provocando l'ennesima tragedia: un furgone è stato travolto da una frana, con il pesante bilancio di due morti e cinque feriti. Inoltre, come si evince anche dai contenuti dell'ultimo rapporto della Commissione antimafia e dalle denunce dei sindacati e delle imprese, le richieste di estorsioni, le frequenti frodi d'identità e le intimidazioni delle organizzazioni criminali sono diventate soffocanti, al punto che molte ditte impegnate nei lavori sull'A3 e in altre grandi opere pubbliche hanno manifestato l'intenzione di interrompere i lavori ed abbandonare i cantieri. Chiedo quindi al Governo quali provvedimenti saranno adottati al fine di realizzare un piano organico di prevenzione ambientale, teso alla corretta e tempestiva realizzazione delle opere relative all'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria; chiedo inoltre quali provvedimenti di carattere eccezionale intende adottare

Signor Presidente, onorevole Ministro, nell'attuale momento di crisi economica e di limitazione delle risorse pubbliche, l'applicazione delle procedure di *project financing* per la realizzazione delle infrastrutture viarie rappresenta una risorsa importante per l'ammodernamento della dotazione infrastrutturale del Paese e per la copertura finanziaria delle dovute operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria, indispensabili ai fini della sicurezza stradale. Al Nord, grandi opere e intere autostrade sono state finanziate dai privati. Vedi, ad esempio, la BreBeMi, finanziata interamente dai privati senza appesantire il bilancio dello Stato e nell'interesse della collettività. Autostrade come la Salerno-Reggio Calabria sono state finanziate non solo con le ordinarie risorse dell'ANAS, ma anche con finanziamenti straordinari per fronteggiare periodici problemi di mobilità e sicurezza. Ciò perché l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, la Catania-Palermo ed altre autostrade meridionali non sono sottoposte a pedaggio e pertanto i costi di realizzazione, gestione e manutenzione di tali autostrade sono interamente interamente a carico dell'ANAS e delle risorse statali, non potendo applicare su tali strade le procedure innovative del *project financing*. La prima domanda che rivolgo al Ministro è se non ritenga opportuno assoggettare a pedaggio l'autostrada Salerno-Reggio Calabria per garantire le occorrenti risorse finanziarie per una gestione moderna e coerente agli avanzati schemi di sicurezza e mobilità già adottati per le autostrade del Nord. secondo luogo, l'apertura ai privati, quando è correttamente disciplinata dalla legge, a garanzia della trasparenza e della concorrenzialità, offre un'implementazione degli investimenti per la realizzazione di opere di interesse collettivo senza accrescere i rischi di infiltrazioni mafiose negli appalti. La lunga storia della Salerno-Reggio Calabria e i sequestri dei cantieri avvenuti nel corso degli ultimi anni testimoniano il contrario. Come emerso dalla relazione annuale sulla 'ndrangheta della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, la costruzione della strada «fu segnata, fin dalle prime fasi, dalla presenza delle organizzazioni mafiose e dal loro intervento, che ne hanno accompagnato la storia infinita fino ai nostri giorni»;

Signor Presidente, signor Ministro, come accade quasi ogni anno, affrontiamo un argomento cosiddetto eccezionale, ma è evidente che quando un evento del genere si verifica puntualmente ogni anno, vuol dire che è diventato ordinario e non è più eccezionale. Sappiamo peraltro benissimo che, secondo la scienza e le attuali conoscenze, gli eventi possono considerarsi eccezionali quando hanno un indice di possibile reiterazione superiore ai cento anni. Quello che sta accadendo e che è accaduto in Calabria è un fatto che invece accade regolarmente: le piogge torrenziali sono un fatto normale; ciò che non è normale è la conseguenza di questi eventi torrenziali che, sia pur ingenti, appartengono alla normalità. Sappiamo anche che il 68 per cento dei Comuni calabresi è considerato a rischio idrogeologico.

Si dice che le condizioni di quell'arteria sono tali perché non si paga il pedaggio; ora noi non vorremmo che il pagamento del pedaggio sia equivalente di sicurezza; che, laddove non si paga il pedaggio, vi sia minore sicurezza; che un costone di una montagna possa franare su un'arteria e che questo possa essere ritenuto accettabile soltanto perché non si paga il pedaggio. Io chiedo quando queste situazioni eccezionali possono rientrare nell'alveo della normalità ed essere affrontate, quindi, con razionalità e con un programma che riguardi il territorio ed il rischio idrologico, che sicuramente affligge la Calabria.

torna ciclicamente agli onori della cronaca, anche recentemente per le tragiche vicende delle morti dovute all'ultima frana. Credo che queste evenienze, al di là della circostanza che ovviamente la competenza del ministro Matteoli non attiene alla materia della Protezione civile, comunque sollevino almeno tre quesiti che mi sembrano utili a fare chiarezza, si spera una volta per tutte, su questa grande opera. La prima questione, che anche altri colleghi hanno sollevato, riguarda la circostanza che sono dati che provengono da una relazione dell'ANAS alla Commissione parlamentare antimafia, così come emersa dai giornali - almeno due volte al mese le imprese che lavorano sulla Salerno-Reggio Calabria subiscono attentati ed intimidazioni.

nella esecuzione del contratto dei lavori. L'ultima questione che emerge, sulla quale chiediamo una risposta, riguarda la copertura finanziaria di quest'opera e i suoi tempi di ultimazione. Il CIPE, nel mese di dicembre, ha deliberato un piano di grandi infrastrutture ma, nell'ambito delle

Signor Presidente, i colleghi senatori che sono intervenuti hanno posto una serie di quesiti cui spero di poter rispondere esaurientemente. Come è a tutti noto,

alla rimozione delle situazioni di pericolo legate agli eventi delle ultime settimane. per l'emergenza, con il compito, tra l'altro, di predisporre un piano generale di interventi. Inoltre, c'è stato un primo stanziamento di 15 milioni di euro per gli interventi urgenti a carico del Fondo della protezione civile, che sarà integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tale stanziamento si va a sommare alla quota parte di 100 milioni di euro destinati alla Calabria per gli eventi atmosferici dello scorso mese di dicembre. L'ordinanza, tra l'altro, si propone la promozione di un processo virtuoso di mitigazione della vulnerabilità e del rischio già presenti sui territori regionali e solo aggravati o resi manifesti dai recenti

posto un rimedio per il ricorso ad interventi di somma urgenza, ai quali seguiranno gli altri interventi urgenti di completamento. In altri tratti, in numero peraltro esiguo, le interruzioni sono state causate dallo slittamento di scarpate sul piano viabile. Tre sono le arterie di competenza statale coinvolte: la strada statale n. 18, la strada statale n. 107 e la strada statale n. 106. L'emergenza è stata fronteggiata dall'ANAS nella seguente maniera: sono stati attivati nove interventi di somma urgenza, finalizzati alla riapertura dell'autostrada, sia pure con limitazioni e scambi di carreggiata. Gli interventi hanno consentito l'apertura dell'autostrada in due fasi: nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, per la tratta Rogliano‑Cosenza e, nella notte tra il 9 e il 10 febbraio, in doppio senso di circolazione sulla carreggiata nord, per il restante tratto San Mango‑Rogliano. Sono state mobilitate dieci imprese con turni di lavoratori anche notturni; sono stati individuati interventi urgenti di completamento delle somme urgenze con la redazione di perizie di completamento per la bonifica; è stata infine effettuata un'analisi globale delle criticità

dei danni, risultano complessi e di notevole proporzione: il loro ammontare economico si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Per quanto concerne la programmazione di interventi di difesa del territorio, la situazione di rischio idrologico nella Regione Calabria può essere riassunta con dati riportati dal piano stralcio per l'assetto idrogeologico

Presidente, mi ritengo soddisfatto della risposta del Ministro, in particolare relativamente all'esigenza del pedaggiamento a valle di un completamento complessivo delle opere di cui oggi iniziamo ragionevolmente a vedere

spostamento delle merci e il commercio. Credo che si debba fare di più affinché queste opere vengano realizzate. Quando poi si parla di rischio idrogeologico, Ministro,

mi rendo anche conto di come, nel corso degli anni, i costi sopportati per sopperire ai danni determinati dai disastri o dagli eventi alluvionali

La tutela dell'ambiente e quindi la difesa dal rischio idrogeologico non dovrebbe essere il primo intervento strutturale sul quale il nostro Paese è chiamato a scommettere?

Presidente, signor Ministro, il decreto anticrisi ha previsto 65 milioni di euro di intervento per gli anni 2009, 2010 e 2011 2010 e 2011 per accompagnare le procedure di privatizzazione della società Tirrenia e consentire la stipula della nuova convenzione che assicura i collegamenti marittimi essenziali. La Tirrenia è uno dei patrimoni importanti di questo Paese, che ha assicurato i servizi di continuità territoriale e di collegamento anche in condizioni difficili, di debolezza strutturale,

Nello stesso tempo, essa ha garantito una quantità di occupazione piuttosto importante. Sotto questo profilo, quindi, la Tirrenia è stata nella storia di questo Paese un patrimonio importante. La procedura di privatizzazione rischia, all'interno delle regole in cui occorre muoversi e se non opportunamente gestita, di creare un momento di difficoltà di creare un momento di difficoltà proprio alle situazioni più deboli, cioè a quei collegamenti più difficili da sostenere sotto il profilo economico e, in generale, alla Come intende il Governo seguire queste procedure procedure in maniera tale da riuscire poi, alla fine, a difendere questi aspetti che, da un lato, sono gli aspetti più qualificanti dell'intervento della società e, dall'altro, sono le situazioni le situazioni economicamente meno sostenibili? Questo è il punto di preoccupazione che è emerso nel dibattito sulla privatizzazione della Tirrenia.

Signor Presidente, onorevole ministro Matteoli, il problema che il Governo ha di fronte, ormai da dieci mesi, con la compagnia di navigazione Tirrenia è noto e semplice nella sua rappresentazione; lo è molto meno per come affrontarlo e condurlo a soluzione. Il tema è quello della liberalizzazione del comparto del cabotaggio marittimo e della privatizzazione della compagnia di navigazione statale Tirrenia. La privatizzazione della compagnia senza la liberalizzazione del settore comporta, come ben evidente, rilevanti fattori di rischio per la collettività. Contrariamente alle dichiarazioni di principio, che in questi casi si sprecano, spesso privatizzare senza liberalizzare significa sostituire un monopolio pubblico con un monopolio privato, con la differenza che con il primo si può avere almeno l'illusione, ogni tanto, di cambiare le cose cambiandone i vertici; con il secondo tipo di monopolio, invece, spesso non si riesce neppure ad avere un interlocutore di riferimento per reclamare per i disservizi. La compagnia Tirrenia, come veniva ricordato, è una compagnia statale con società regionali ad essa collegate, avente condizioni e caratteristiche di servizio tra loro differenziate. Ciascuna, accomunata dalla necessità di garantire il mantenimento dei servizi universali di continuità territoriale, costituiti da collegamenti con le piccole isole: dall'arcipelago delle Eolie, dove proprio nei giorni scorsi abbiamo assistito a vibranti manifestazioni di protesta, ai collegamenti con la nostra piccola isola di Capraia. Da tempo le è stato presentato, signor Ministro, il piano industriale da parte della compagnia Tirrenia che prevede, con l'accordo di tutte le organizzazioni sindacali, la riduzione dei costi di gestione, nell'ordine del 23 per cento, unitamente alla privatizzazione della stessa compagnia. Le chiediamo, signor Ministro, quali sono le sue valutazioni circa l'auspicabile spacchettamento della Tirrenia in società regionali: secondo lei, è da realizzare nella fase di privatizzazione o successivamente ad essa? Oppure non è da farne niente? da farne niente? Signor Ministro, quali garanzie, inoltre, il suo Ministero e il Governo intendono offrire alla conoscenza del Parlamento e dei cittadini sul mantenimento dei servizi universali di collegamento territoriale con le piccole isole? servizi per i quali (è bene ricordarlo ed è noto), indipendentemente dalla natura del soggetto gestore, occorrono contributi di sostegno da parte dello Stato. Signor Presidente, onorevole Ministro,

società. Sintetizzando, gradiremmo quindi sapere qual è la posizione del Ministro rispetto alle procedure per quanto riguarda la privatizzazione della società e anche ai disservizi che si stanno verificando a danno dei cittadini interessati all'utilizzo delle navi della Tirrenia per tratte minori.

gli italiani ci rimettono 15 euro. La Tirrenia sembra una barca piena di falle che perde 200 milioni l'anno, ma i compensi dei consiglieri e dei sindaci si sarebbero addirittura triplicati con un aumento da 320.000 euro nel 2003 a 973.531 nel 2007, senza considerare Il gruppo ha ricevuto dal 2003 al 2007 contributi statali in conto esercizio per 1,24 miliardi di euro. euro. L'amministratore delegato Franco Pecorini è alla guida della compagnia dal 1984, un *manager* inamovibile che ha resistito a diciassette

forse con gli stessi metodi di Alitalia, utilizzando, cioè, la socializzazione delle perdite e la privatizzazione dei profitti? Forse, come per Alitalia, le passività potranno confluire in una *bad* *company* e le attività in una *good* *company*. L'Italia dei Valori è molto preoccupata sia per il taglio alle rotte, per la qualità dei servizi erogati soprattutto nelle piccole isole e per i loro collegamenti, sia per una privatizzazione molto discutibile che potrebbe, signor Ministro, portare a

Signor Presidente, signor Ministro, dal 6 novembre 2008 si è avviata in maniera più concreta, con una deliberazione del Consiglio dei ministri, la procedura di privatizzazione della fare innanzitutto una premessa. Siamo assolutamente favorevoli alla circostanza che la Tirrenia venga privatizzata e che si operi finalmente una razionalizzazione economica e finanziaria di questa società,

con riferimento ad esempio ai collegamenti con le isole minori, significa garanzia della parità di trattamento tra cittadini, indipendentemente dal territorio nel quale si trovino. Pertanto, la continuità territoriale non può essere interpretata in senso minimalistico in una procedura di privatizzazione:

fruizione turistica di quelle isole nei periodi estivi e destagionalizzati. Tutto ciò non sembra essere avvenuto. Da allora c'è un *can-can* di

garantisce anche il collegamento Eolie-Napoli, che è una linea fortemente produttiva per il territorio eoliano. In secondo luogo, si tratta che cosa si intende fare dell'eventuale scorporo della società Siremar dalla Tirrenia per garantire impulso a questa società regionale, soprattutto per l'importanza che essa ha con riferimento alle isole minori. Infine, vorremmo sapere se è stata affrontata seriamente, in sede europea, la questione della deroga per lo scorporo della Siremar dalla

Comprendiamo che la privatizzazione della Tirrenia sia obbligata dalle prescrizioni comunitarie e che possa essere un'opportunità per garantire maggiore efficienza nei collegamenti. In modo particolare, il tema che mi che mi impegna è quello dei collegamenti con le isole minori che, per la Regione Siciliana, sono molto rilevanti, non solo dal punto di vista sociale, ma anche per gli interessi economici che esse rappresentano e che possono essere ulteriormente sviluppati da una politica turistica che non può prescindere

Abbiamo poco tempo: la proroga concessa scade alla fine di quest'anno e rischiamo effetti gravissimi perché l'allarme è rilevantissimo. Signor Ministro, avendo apprezzato molto il tono, l'attenzione e la cura con cui lei ha seguito questa vicenda

vi è piena condivisione anche da parte del Ministro dell'economia, che troppo spesso ha attinto a queste risorse per ragioni estranee alla loro destinazione: in un caso come questo sarebbe davvero incomprensibile che frapponesse ostacoli all'impiego necessario delle stesse risorse. Ma il tema è più ampio e riguarda le società regionali. La Regione Siciliana non è contraria all'assunzione piena di responsabilità in capo alla Siremar, ma non riesce da tempo ad accedere ad una *due diligence* che consenta di verificare il patrimonio, la dotazione organica, i mezzi bilanci di questa società. È una condizione che rende impraticabile anche la più ampia buona volontà per corrispondere ad una indicazione del Governo che può trovare una soluzione positiva. PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere congiuntamente agli interroganti il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Matteoli.

prima di ogni altra cosa, voglio fare una precisazione che riguarda i collegamenti con le isole minori in Sicilia, in risposta alle voci di presunti tagli che hanno avuto come conseguenza le giuste proteste dei residenti. Come già ho avuto modo di chiarire, non ho disposto alcun taglio di risorse, né alcuna soppressione dei collegamenti marittimi tra la Sicilia e le sue isole minori. In verità, in data 9 gennaio, dopo un incontro con l'assessore Bufardeci e i sindaci dei Comuni isolani interessati, ho inviato una lettera a Tirrenia e a Siremar dando precise direttive sul mantenimento dei collegamenti. Questa è la realtà. Basta che un giornale scriva mezza frase e ci sono coloro che si mettono a dieta ‑ come qualcuno in maniera ironica ha detto - e nascono proteste, ma la verità è questa che ho avuto modo di dire; non c'è nulla di diverso da questo.

il processo di privatizzazione prende avvio con la legge n. 296 del 2006 (la finanziaria del e prevede, al fine di completare il processo di liberalizzazione del cabotaggio marittimo e di privatizzare le società esercenti i collegamenti marittimi con le isole maggiori e minori, la stipula di nuove convenzioni con dette società entro il 30 giugno 2007 con scadenza non anteriore

erano scadute le convenzioni. E come ha ritenuto di comportarsi il Ministro? Si è recato più volte in Europa. I sindacati mi invitavano a chiedere una proroga di quattro anni; l'Europa ci offriva sei mesi di proroga

Aggiungo che con delibera del CIPE del 9 novembre 2007, n. 111, si è provveduto a determinare sia i criteri per l'individuazione delle rotte di servizio pubblico che quelli per individuare la giusta compensazione per tali servizi.

57, ha assegnato alle Regioni interessate le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione dei servizi di cabotaggio marittimo di interesse pubblico da svolgere all'interno di una singola Regione e al successivo comma 3 ha previsto il passaggio a titolo gratuito dei pacchetti azionari delle società regionali dal gruppo Tirrenia alle Regioni che ne avrebbero fatto espressamente richiesta.

Inoltre, il successivo decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto l'erogazione di risorse aggiuntive e fissato per il corrente esercizio una dotazione di bilancio pari a 174 milioni di euro allo scopo di consentire l'attivazione della procedura di privatizzazione del gruppo Tirrenia. a questa cifra, per poter mantenere i collegamenti con le isole minori, vi è la necessità di trovare 46 milioni di euro. è un tavolo aperto di consultazione. Ci sono stati fino ad ora tavoli di consultazione tra il Ministero e le singole Regioni interessate. La prossima settimana ci sarà, invece, un tavolo dove saranno chiamate ovviamente le Regioni, sarà chiamata la Tirrenia e naturalmente, in quella occasione, cercheremo di trovare le soluzioni indispensabili.

me, senatore Filippi, lei conosce il nostro arcipelago e sappiamo tutti, per esempio, che vi è un traghetto che tutti i sabato mattina parte da Capraia per arrivare a Livorno con un solo passeggero. È chiaro però che nel bando di gara che andremo a fare non potremo consentire che il privato che andrà a rilevare Tirrenia si prenda solo la parte buona e scarichi la parte meno buona, perché faremo un bando dove

è un peso economico, durante il periodo estivo queste isole rappresentano una ricchezza per il Paese e quindi non possiamo certamente abbandonarle.

La Commissione europea, in risposta a quanto richiesto dall'Italia, in data 19 dicembre 2008, ha chiesto elementi aggiuntivi in merito all'intera procedura di privatizzazione con particolare riferimento alla definizione delle rotte di continuità territoriale e alle fasi di privatizzazione, chiedendo sostanzialmente di poter condividere un percorso prestabilito con tempi e fasi definitive. La Commissione, in particolare, nel sottolineare La proposta italiana presentata alla Commissione dell'Unione europea, in linea con quanto previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 207, è stata quella di procedere alla privatizzazione del gruppo entro il 31 per avviare dal 1° gennaio 2010 le nuove convenzioni per consentire alla nuova proprietà del gruppo di assestarsi e rendere competitivo il servizio offerto e successivamente procedere alla liberalizzazione dell'intero settore, così come previsto dal regolamento (CEE)

esaurito l'argomento. D'altra parte, la sua idea di approfondire in Commissione tutti gli aspetti di questa vicenda, che indubbiamente è ai suoi prodromi e che sarà di enorme complessità, mi sembra vada accolta. Quindi, accogliamo con soddisfazione l'idea di approfondire e di accompagnare *l'iter* di privatizzazione della Tirrenia attraverso un approfondimento nella sede competente, l'8a Commissione permanente del

Infatti, un conto sono le sue rassicuranti dichiarazioni su ciò che non ha fatto, cioè disposizione di tagli, altro ciò che purtroppo ha fatto il suo collega Tremonti non rifinanziando il dovuto.

difficile, che vive realtà come quelle delle nostre isole. È stato spesso evocato anche in quest'Aula lo spettro di Alitalia;

Tuttavia, non posso considerarmi soddisfatto su alcune precise domande che l'Italia dei Valori le ha rivolto in merito alla gestione molto disinvolta del *management* della Tirrenia, sulle consulenze e sui compensi. Per questa ragione,

Signor Presidente, signor Ministro, anche noi, come lei, riteniamo che questo sia un tema che non possa esaurirsi in un *question time* di qualche minuto. Per la verità, noi abbiamo presentato una mozione, il 20 novembre 2008, proprio su questo tema e credo che, al di là dell'utile audizione che lei

noi abbiamo ad oggi solo una certezza: la proroga comunitaria del servizio fino a tutto l'anno 2009; ha poi parlato della possibilità di reperire - perché ancora oggi non vi è certezza - i 46 milioni di euro che sono necessari per garantire il servizio in quest'anno; ha detto che non vi è alcuna intenzione di procedere allo scorporo della SIREMAR dalla Tirrenia e che non vi è alcuna intenzione di assumere un'iniziativa in sede europea perché questo possa avvenire ovvero vi possano

ribadisco volentieri il mio apprezzamento per lo stile e la sensibilità con la quale lei sta seguendo questa vicenda, che è delicata e rimane ovviamente aperta.

credo che in una sede più attenta come la Commissione competente potremo approfondire alcune opportunità rispetto alle esperienze già fatte dalla Regione Siciliana, che ha provveduto per una parte ad assicurare servizi aggiuntivi a mezzo gara perché essa possa misurarsi, d'accordo con il Governo, con una gestione il più autonoma possibile del collegamento con le isole minori, che sono non solo una responsabilità che attiene al Governo regionale, ma anche una grande opportunità per quello che esse rappresentano. Credo che una riflessione una riflessione *bipartisan*, di tipo istituzionale, possa consentire di individuare quanto meno con la Regione Siciliana delle soluzioni più avanzate, certo rispettose delle prescrizioni europee che, come hanno imposto la privatizzazione, impongono anche una gara unica che indubbiamente irrigidisce il procedimento e rischia di non definire soluzioni più flessibili, come casi come questo forse richiederebbero, trattandosi di condizioni oggettivamente diverse nel territorio nazionale. *(PdL)*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, lo scorso 11 febbraio il Senato della Repubblica ha licenziato con voto di fiducia il decreto‑legge cosiddetto tra le misure in esso contenute destano forte preoccupazione le nuove regole introdotte per il così detto noleggio con conducente. In particolare, dette nuove regole prevedono l'obbligo di rientro nella rimessa dopo ogni singolo servizio; divieto di sosta in luogo pubblico anche durante il servizio; la compilazione di autocertificazione per ogni entrata. Tali nuove regole modificano di fatto le norme previste dalla legge n. 21 del 1992 («Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea») e penalizzano sostanzialmente l'attività di noleggio con conducente. Preso atto che l'approvazione delle sopra riportate norme ha creato grande allarme e preoccupazione tra le associazioni di categoria, che vedono oltremodo penalizzata la propria attività lavorativa e minacciano

stante il momento di crisi che attanaglia tutti i settori. Chiedo, pertanto, al signor Ministro se ritenga di dover intervenire in tempi brevissimi, nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni, pur nella doverosa salvaguardia della distinzione degli NCC dal servizio taxi, al fine di riportare i cosiddetti NCC nell'alveo delle norme previste dalla legge n. 21 del 1992 o, in subordine, se ritenga di dover concordare eventuali modifiche alla predetta legge dopo un confronto con le associazioni di categoria. signor Ministro, nel decreto milleproroghe recentemente approvato da questo ramo del Parlamento senza

con questa modifica di legge si introducono vincoli assai stringenti per quanto concerne, in particolare, l'accesso ai territori dei Comuni, segnalando che la disposizione interviene in modo dettagliato in una materia nella quale non è prevista una competenza legislativa statale, ostacolando il

Ministro: cosa intende fare il Governo per non allarmare e aggravare ulteriormente lo stato di difficoltà di questa categoria? Vorrei sapere se ritiene che questo sia il modo corretto per legiferare su una materia che riguarda 200.000 cittadini e poi, siccome abbiamo notizia che in un incontro con le categorie lei ha assicurato un intervento rapido del Governo per risolvere il problema, se questo intervento c'è, se sarà per decreto e cosa succederà nei prossimi giorni. Le chiediamo in quest'Aula, che non ha potuto discutere questo provvedimento, di essere particolarmente preciso, in nome dei 200.000 lavoratori di questo settore, che sono in grave allarme in una situazione economica particolarmente difficile.

questo emendamento, che ha creato non solo difficoltà, ma anche un grave allarme per quanto riguarda gli NCC.

con conducente a chiamata diretta, per un particolare servizio personalizzato, mentre il taxi è un servizio a chiamata numerica per il trasporto di persone abilitato a servizio pubblico. Ci sono state proteste da parte di questi noleggiatori che possono essere condivise. Signor Ministro, non vorrei che l'attuale maggioranza

trasporti*. Proprio ieri, 18 febbraio, ho tenuto un incontro con i rappresentanti sindacali di noleggiatori e tassisti,

dei rappresentanti dei sindacati, perché c'era in ogni intervento che ascoltavo una grande preoccupazione di evitare una guerra che sarebbe, tra l'altro, una guerra tra poveri, tra noleggiatori e tassisti. La prima riunione di questo tavolo tecnico si terrà martedì 3 marzo e, nel frattempo, mi sono impegnato, d'accordo anche con la Presidenza del Consiglio, ad intervenire con gli strumenti che si riterranno più idonei, come sollecitava la senatrice Rizzotti, sulla norma contenuta nel decreto milleproroghe.

A titolo di chiarimento, occorre ricordare anche - qualcuno lo ha già detto - che la materia si qualifica come potestà concorrente ai sensi del titolo V della Costituzione, con la conseguenza che la legislazione statale può intervenire solo per dettare principi di carattere generale, ad esempio disciplina della concorrenza, che salvaguardino l'autonomia di regolamentazione del servizio di trasporto pubblico locale, tant'è che la legge n. 21 del 1992, su cui si va ad incidere, è una legge quadro. È evidente che in tale ottica le modifiche introdotte dal comma 1-*quater* dell'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 parrebbero presentare alcune perplessità, in quanto verrebbero a limitare il diritto della libera circolazione, imponendo obblighi di carattere amministrativo per disciplinare l'esercizio del servizio nel proprio territorio, così come pure obblighi di stazionamento e di documentazione, che esulano dal mero esercizio La predetta normativa parrebbe inoltre porsi in contrasto con la direttiva 123 della Comunità europea del 2006, il cui termine di recepimento scade il 28 dicembre 2009. prevede l'obbligo degli Stati membri di rispettare il diritto dei prestatori di servizio di operare in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno sede e di assicurare il libero accesso dell'attività di servizio sul proprio territorio. La predetta direttiva esclude dal proprio ambito di operatività i trasporti locali ed i taxi ma non il noleggio con conducente che, per le proprie caratteristiche, legate a una maggiore autonomia contrattuale rispetto al settore taxi, sarà oggetto della prescritta liberalizzazione. È vero quanto è stato ricordato da

ma a condizione che si intervenga in un altro provvedimento per annullare l'emendamento che è stato presentato in Senato. Non possiamo non tenere conto di questa condizione

Presidente, apprezzo molto la risposta del Ministro. Sono fiduciosa in un rapido annullamento della suddetta norma, per ridare sostegno e possibilità di operare a una categoria di migliaia di operatori che temono di non poter più provvedere alle loro famiglie, non potendo usufruire di alcun tipo di ammortizzatore sociale nel caso venisse ulteriormente penalizzata la loro attività lavorativa.

prendo per buono l'impegno del Governo di intervenire rapidamente, non appena la legge sia stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*. Vorrei ricordare che, come Partito Democratico, avevamo dato la disponibilità

un intervento veloce. Vogliamo però ricordare che qualcuno nella città di Roma, nella fattispecie il sindaco Alemanno, ha scatenato, in ossequio ad alcuni impegni elettorali, una guerra tra poveri che mette a repentaglio 40.000 imprese e 200.000 famiglie in tutta Italia. quindi che vadano rispettate le leggi, la Costituzione e il suo Titolo V e tutte le normative che ci permettono di costruire un processo legislativo più equo e meglio meditato.

ragioni, signor Ministro, vigileremo su questa vicenda perché si concluda nel modo più celere possibile. Signor Presidente, signor Ministro, anche noi prendiamo atto del suo impegno, delle sue risposte e della necessità che non si scatenino, soprattutto in una fase delicata come questa, guerre tra poveri e tra lavoratori che vedono messo a repentaglio il loro posto di lavoro. Già si tira la cinghia e vogliamo proprio augurarci che da questo tavolo scaturiscano atti concreti, ossia